Ha facoltà di parlare il senatore Lepri per illustrare la mozione n. 34

una mozione per dare voce al grido di dolore, alle lacrime, alla rassegnazione di milioni di persone che vivono oggi nel nostro Paese una condizione di povertà materiale. Non è inutile ricordare che ce ne sono altre di povertà: istituzionali, relazionali, per esempio. Ma oggi vogliamo concentrarci sulle questioni relative alla povertà materiale: una povertà che sta aumentando drammaticamente senza che ci sia una pari crescita di consapevolezza Grazie, Presidente. Sono molti i dati indiscutibili che rappresentano questo drammatico fenomeno. Basti per tutti citare il dato dell'ISTAT che ci riporta come dal 2010 al 2011 la percentuale di persone in condizioni di povertà assoluta sia passata dal 6,9 per cioè 4 persone su 100, dal 2010 al 2011, sono cadute in condizioni di povertà assoluta. Ma ce lo dicono soprattutto coloro che sono in prima linea nel contrasto alla povertà:

ma forse non tutti i colleghi sono a piena conoscenza del fatto che in questo comparto sono stati fatti, nel corso di questi ultimi cinque sei anni, dei tagli draconiani e non i tagli lineari (unica

Pensiamo solo al fatto che qualche anno fa il Fondo per le politiche sociali ammontava a oltre 800 milioni di euro, mentre nel 2012, nel bilancio di previsione 2013, era di 40 milioni.

la totale difficoltà in cui versano i servizi di contrasto alla povertà. anche all'interno della nostra maggioranza vi sono opinioni diverse sul modo in cui contrastare questo drammatico fenomeno.

alle pur importanti ricette della sussidiarietà. Sono proprio le realtà caritative (il volontariato e le imprese sociali) a dirci che occorre intervenire senza altro indugio con più risorse. Altra cosa è invece ritenere che il terzo settore debba e possa intervenire in modo assolutamente attivo, da protagonista, nelle politiche di contrasto al fenomeno.

totale disponibilità di risorse per realizzare la sperimentazione della nuova *social card*; infine, il completamento per tutto il 2013 dell'iniziativa a regime della *social card*, già avviata con il Governo Berlusconi. Il nostro Gruppo interverrà con le parole dei colleghi Favero, Pegorer e D'Adda su altre questioni e, in particolare, sulla morosità incolpevole che riguarda migliaia di persone che rischiano di non poter più abitare in case di edilizia residenziale pubblica a causa - dell'impossibilità di pagare con risorse proprie, dimostrando la loro incolpevolezza e non essendovi più, se non in minima parte, le risorse di cui fino a quest'anno potevano disporre grazie agli interventi regionali e comunali. Non dimentichiamo che qualche anno fa il Governo tagliò in modo definitivo le risorse per finanziare la morosità incolpevole. Ebbene, anche questo fenomeno ormai è insostenibile e sta determinando situazioni davvero drammatiche. In conclusione, noi riteniamo che su questo tema debba esservi un sussulto di responsabilità, una maggiore attenzione da parte del Governo e del Parlamento, ben sapendo che le misure di contrasto debbono fare i conti con l'esigenza di una nuova visione e di una nuova prospettiva; sappiamo tuttavia che oggi le povertà non possono aspettare un ridisegno delle politiche pubbliche e quindi chiediamo subito, al di là degli importi minimi che abbiamo indicato

Signor Presidente, oggi affrontiamo un tema sicuramente centrale, ma in fondo non disgiunto da quello che abbiamo discusso ieri con il Presidente del Consiglio.

la voglia di dire di essere in uno stato di indigenza. Questa è una delle preoccupazioni che dobbiamo affrontare insieme. Oggi prima di tutto, signora Vice Ministro, abbiamo la necessità abbiamo la necessità di ricostruire forse una nuova mappa delle povertà, che ci deve trovare partecipi come attori della politica. È una mappa nuova, perché proprio in queste nuove povertà ci è chi non immaginiamo che in questo momento abbia difficoltà; in essa c'è veramente, come dicevo prima, quel vicino di casa che abbiamo conosciuto e che vediamo tutti i giorni, ma che noi stessi non sappiamo

per tutto quello che riguarda le persone. E le persone non sono lontane o diverse dal mercato, signora Vice Ministro. In questi anni abbiamo anche immaginato, in maniera non sempre facile, che occorresse procedere ad una ricostruzione di piattaforme inalienabili, che non sono semplicemente realtà retoriche o teoriche. Si è infatti ritenuto che, dopo il fallimento di quasi tutte le teorie economiche che ci hanno portato fino ad oggi, con la drammaticità del momento,

importante: come ha detto il collega prima, penso che sia doveroso trovare delle provviste finanziarie da mettere poi a disposizione): dobbiamo recuperare anche quello che c'era prima, uscendo dal virtuale e tornando alle reti sociali, che esistevano. La teoria non ci spiega come funzionavano,

che ci siano aspetti in cui un agente sociale riesce a capire prima di un amministratore dove si deve e si può intervenire. Abbiamo proposto anche che, in questo contesto, si riattivi quello che riteniamo l'aspetto virtuoso del federalismo, non per fare sperequazioni, ma per consentire anzi che alcune situazioni

perché quella sarà forse una parte essenziale della nostra capacità di rispondere nell'immediato. Il Governo, lo Stato, le Regioni possono mettere a disposizione provviste finanziarie e creare le condizioni attraverso politiche attive, ma dobbiamo conoscere la nostra rete sociale. Usciamo un po' dal virtuale, torniamo alla realtà di tutti i giorni, torniamo alla solidarietà di vicinanza e facciamolo con la correttezza che credo possa riunire tutti, al di fuori della connotazione politica, ricordando le nostre grandi tradizioni. Le chiedo, signora Vice Ministro, di apprezzare la nostra mozione,

oggi può essere una giornata bella per il Parlamento, una giornata dove al centro del nostro interesse e della nostra discussione ritorna ad esserci l'ultimo, il più debole: quelli che spesso chiamiamo «gli invisibili». La crisi finanziaria, che da qualche anno si è manifestata in Italia, ma che ha origini mondiali, ha bisogno di una risposta immediata, che nella mozione che illustro definiamo «innovativa e concreta». Si rende necessario, urgente e improcrastinabile un intervento complessivo per riorganizzare il programma del *welfare* italiano, teso a migliorare la vita dei cittadini, nella situazione di difficoltà e di povertà che molti attraversano in questi giorni: non solo, quindi, una risposta finanziaria, ma culturale, sociale e politica. Assistiamo inermi, in questo periodo, alla trasformazione della povertà in miseria e questo impoverimento sta producendo una caduta dei consumi vertiginosa e l'aumento a dismisura della disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Questa nuova povertà provoca una nuova vulnerabilità sociale: la persona lasciata sola, sopratutto in contesti urbani difficili, fatti di relazioni deboli, diventa sempre più fragile, con una vita sociale disarticolata, rendendo la vita quotidiana più ricattabile dagli insostenibili aumenti di tariffe e di servizi a pagamento. Ciò coinvolge molte famiglie e le casse degli enti locali-territoriali sono spesso in difficoltà per dare le risposte necessarie alle esigenze di tutti noi cittadini. E allo Stato impossibilitato a svolgere il suo ruolo sociale, ringraziando Iddio, si è aggiunto e, non di rado, sostituito, l'associazionismo del *non profit*. La situazione finanziaria, dei consumi e il deterioramento dello Stato sociale e dei beni primari sta peggiorando dai dati Istat del maggio 2013, riferiti al 2011 e al 2012, dalla Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dai dati dell'Unione europea dello stesso mese emerge che la deprivazione materiale interessa non solo i cittadini con i redditi più bassi ma anche coloro che dispongono di redditi mediamente più elevati.

nel 2012, in Italia, 1.822 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti, hanno vissuto in condizione di povertà relativa, mentre il 7 per cento, pari a 723.000 minori, ha vissuto in condizioni di povertà assoluta. La quota è stata maggiore nel Mezzogiorno, pari al 10,9 per cento, rispetto al 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese. I dati forniti da Confcommercio confermano che il continuo deteriorarsi del reddito e dell'occupazione ha portato nel 2013 a una contrazione della domanda ancora più negativa rispetto al 2012, mentre la contrazione dei consumi nel biennio 2012-2013 risulta pari al 7,3 per cento, percentuale che equivale ad una diminuzione della spesa delle famiglie di circa 52 miliardi di euro.

L'Eurostat conferma questo dato in maniera visiva, posizionando l'Italia al quarto posto tra i Paesi d'Europa, dopo Grecia, Spagna e Portogallo, per i dati aggregati della disoccupazione giovanile. Alla disoccupazione giovanile va aggiunto il dato negativo della contrazione degli occupati cosiddetti adulti, con l'espulsione dal mondo del lavoro di cittadini che hanno difficoltà alla ricollocazione in nuovi lavori o aziende, sia per un fattore d'età che per specializzazione. Si è registrato fra il 2011 e il 2012 circa un milione di occupati in meno solo nel settore cosiddetto degli adulti. Sempre di più le persone che sono considerate i poveri di oggi fino a qualche anno fa erano considerati la nostra classe media che riusciva ad arrivare, con un'espressione felice, «a fine mese» dignitosamente. Oggi queste persone ricorrono sempre più alle mense dei poveri per sopravvivere. Colleghi, il nostro impegno dovrà essere volto a rafforzare il rapporto tra il Parlamento, il Governo e le forze sociali per combattere tutti insieme, anche insieme alle associazioni *non profit*, l'emergenza della povertà, stabilendo di restituire dignità alla persona, alla famiglia e al lavoro di tutti: un percorso comune sulle modalità e sui tempi di soluzione. Chiediamo nella nostra mozione di riferire annualmente al Parlamento le misure e le iniziative che si intendono attuare contro la povertà, non solo a sostegno del reddito, ma principalmente in termini di servizi erogati alle famiglie, a partire dalla scolarità fino ai trasporti pubblici, valorizzando sussidiariamente gli enti locali e le organizzazioni non profittevoli. Dobbiamo invertire la tendenza dei tagli lineari nell'assistenza e nei servizi di base ai cittadini e dobbiamo aggredire, invece, la spesa pubblica improduttiva, legando la spesa alla responsabilizzazione dei centri erogatori. Poi dobbiamo impegnarci nel promuovere un'integrazione reale e vera tra le politiche socio-assistenziali e sanitarie; dal loro giusto equilibrio potremmo avere i risultati nel medio periodo. dobbiamo rilanciare il Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, denominato «Aiuta l'Italia che aiuta». Tale piano, promosso dal Governo Berlusconi IV, ha dato ottimi risultati in termini di risposta alle esigenze dei cittadini. rimettere in pista gli strumenti contemplati da quell'esperienza, quale ad esempio la *social card*, che ha dato dei risultati immediati: uno strumento che comunque va utilizzato in chiave sussidiaria delegando le associazioni *non profit* alla sua gestione. alla conclusione, il mio invito, espresso anche nella mozione, è a trovare in quest'Aula e nel Paese una sintesi e una convergenza sul problema che non dovrebbe dividerci né sull'analisi né sulla soluzione. Il dolore di questi mesi, le morti della disperazione, la miseria che sempre di più è presente nella nostra vita e nelle nostre città ci deve spingere a moltiplicare gli sforzi di unità e di soluzione, per un Paese più moderno che rispetta gli individui e accompagna la famiglia nel percorso della vita.

Signor Presidente, signora Vice Ministro, i rapporti economici continuano a fotografare un'Italia in piena crisi: i dati sull'inattività e sull'occupazione sono tra i peggiori d'Europa. Secondo i dati ISTAT aggiornati a marzo 2013, l'occupazione su base annua diminuisce dell'1 per cento e il tasso di disoccupazione si attesta al 12,8

Secondo il rapporto di Confcommercio, «L'economia e il lavoro dentro la crisi», presentato il 22 marzo scorso, nel 2013 in Italia ci saranno oltre 4 milioni di poveri e una compressione dei consumi del 2,4 per cento. Sono più di 9 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito e quindi a rischio di povertà ed esclusione sociale. sono disoccupati e inoccupati, cittadini che non riescono più a trovare lavoro, che non lo cercano, che hanno perso la speranza. Sono cittadini che hanno perso la motivazione; sono cittadini disperati; sono cittadini che hanno bisogno che lo Stato li accompagni nel loro progetto di vita, che faccia credere loro di poter avere un futuro. Come sottolineato da Codacons, la diminuzione dei consumi interessa in modo drammatico quelli alimentari, scesi del 4,7 per cento rispetto al febbraio 2012. Secondo i dati forniti dal rapporto «Reddito e condizioni di vita» dell'ISTAT, il 28,4 per cento delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, per la Strategia Europa 2020: aiutare le persone a rischio di povertà, incrementare il tasso di occupazione, tutelare i cittadini italiani che non riescono più a vivere. Nel rapporto diffuso nell'ottobre 2012, la Caritas evidenzia come tra le persone che si sono rivolte ai suoi centri nel 2011 vi sia un aumento di quelle appartenenti a categorie che sino a poco tempo fa non erano interessate

e una parte addirittura una pensione al di sotto dei 500 euro al mese. Io vivo in una città della Sicilia, Catania. Ebbene, è una cosa che mi ha stupito molto, colleghi,

Noi abbiamo una grande responsabilità: non si può permettere che un uomo o una donna che hanno vissuto la propria vita nella nostra terra siano costretti a perdere la dignità sancita dall'articolo 3 della Costituzione italiana e a dover andare a raccogliere i rifiuti per poter vivere.

e, nonostante ne siano stati ad oggi salvaguardati circa 130.000, il fenomeno resta comunque di dimensioni drammatiche. Ci sono ancora 111.000 lavoratori che sono a rischio di perdita di lavoro. Questo avviene oggi. Dobbiamo trovare il modo di aiutare i cittadini a vivere una vita dignitosa. politiche intraprese fino ad oggi per sconfiggere la povertà, come il *bonus* gas*,* il *bonus* energia, i contributi per gli affitti e i vari assegni, è mancato un disegno organico di integrazione al reddito. al reddito. Anche la sperimentazione della *social* *card* appare una misura debole e, come diceva ieri la senatrice Sara Paglini, è una misura che toglie dignità al cittadino. Non dobbiamo fare l'elemosina ai cittadini. Siamo cittadini con pari dignità, tutti. A fronte di un quadro così drammatico, sarebbe necessario, è necessario avviare una politica di lotta alla povertà, che riprenda gli esempi migliori europei. L'Italia è l'unica nazione anzi, non l'unica: c'è la Grecia insieme a noi - a non aver istituito un reddito di base, un reddito minimo di cittadinanza, un reddito di dignità: perché di questo stiamo parlando. Siamo gli unici in Europa. Il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, con 540 voti a favore a fronte di 30 contrari. Tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema, adottata nel 2008, ha sancito in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione europea - e quindi anche dell'Italia e delle persone che vi risiedono stabilmente ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale. In attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale - colleghi, fondamentale destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica». La piena partecipazione alla vita sociale è richiesta, come obiettivo da garantire dalla Repubblica italiana, dall'articolo 3 della Costituzione. Misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti in tutta Europa. Il reddito di cittadinanza è lo strumento che assicura, in via principale, l'autonomia delle persone e la loro dignità. Il reddito di cittadinanza è l'unico strumento che garantisce la flessibilità del lavoro, perché, se collegato a una vera riforma del *welfare* italiano, a una riforma dei servizi pubblici italiani, alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici se collegato al sistema nazionale della certificazione delle competenze del cittadino, garantisce allo Stato, al cittadino, alle aziende la possibilità di riprendersi dalla crisi.

il reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero dei cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. di procedere al riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali concordato in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di rendere queste risorse immediatamente disponibili alle Regioni stesse e, quindi, agli enti gestori; di reperire le risorse necessarie, anche attraverso la lotta all'evasione fiscale e la redistribuzione delle retribuzioni, oltre che delle pensioni;

dopo la votazione delle mozioni sulle politiche di contrasto alla povertà si passerà alla votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico per l'elezione di nove componenti effettivi e di nove supplenti della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

i documenti al nostro esame ci richiamano con forza a porre l'attenzione sul tema di una crescente povertà quale possibile campanello d'allarme dell'insorgere di una grave crisi sociale nel nostro Paese. Ieri lo stesso presidente Letta, qui nell'Aula del Senato, nel corso del suo intervento di replica al dibattito sul prossimo Consiglio europeo, ci ha ricordato che: «Come «Come frequentemente capita nelle società occidentali, chi è in condizioni di povertà estrema spesso e volentieri non è cittadino dell'arena politica». Nell'affrontare la questione della povertà in Italia - lo ricordava chi mi ha preceduto - occorre sicuramente partire dai drammatici dati dell'ISTAT che evidenziano come, alla fine del 2012, fossero quasi 15 milioni gli individui in condizione di deprivazione o disagio economico:

La presa d'atto di questa situazione, confermata dai dati di Confcommercio, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della Caritas e dell'Eurispes, deve farci riflettere sulle cause profonde di questo fenomeno, che non accenna a diminuire, ma che potrebbe ulteriormente aggravarsi senza precisi interventi correttivi nelle politiche redistributive. Da questo punto di vista, sono stati sicuramente importanti gli interventi normativi che hanno portato all'aumento del Fondo nazionale per le politiche sociali di 300 milioni di euro, attuati dall'ultima legge di stabilità, e alla stessa sperimentazione della nuova *social card.* risulta difficile pensare di superare questa drammatica situazione senza comprendere le ragioni ad essa sottese, ragioni molto profonde e indicative di una vera e propria crisi di sistema. L'Italia - lo ricordava ancora chi mi ha preceduto - è, insieme alla Grecia, l'unico Paese europeo dove ancora non esistono una politica unitaria di lotta alla povertà e un'ultima rete di protezione sociale per le famiglie al di sotto di una determinata condizione economica. Com'è noto, il premio Nobel Joseph Stiglitz sostiene che, quando le disuguaglianze crescono, s'innesca una spirale negativa, egli altresì rileva che, nei Paesi dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, il prodotto interno lordo tende a Sempre secondo l'analisi di Stiglitz e dello stesso Krugman, il problema principale di tutte le economie avanzate e altamente industrializzate è rappresentato dalla debolezza della domanda aggregata, cioè la domanda di beni e servizi espressa da un sistema economico nel suo complesso. Tenuto conto poi del fatto che la porzione di reddito spesa per l'acquisto dei beni e servizi è, per forza di cose, maggiore nei redditi bassi, la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi è diventata un problema strutturale. Se far ripartire i consumi è fondamentale per far ripartire l'economia, ben si comprende dunque l'importanza di adottare politiche che favoriscano una più equa distribuzione della ricchezza. Da un recente studio commissionato dalla UE nell'ambito del Settimo Programma quadro a un *pool* di gruppi di ricerca di diverse università europee emerge che l'Italia è tra i Paesi che registrano le maggiori disuguaglianze nella distribuzione dei redditi, seconda solo al Regno Unito nell'Unione europea e con livelli di disparità superiori alla media dei Paesi OCSE. Sempre da questo studio, emerge, inoltre, che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e che la ricchezza si sposta sempre più verso la popolazione anziana, a scapito delle giovani generazioni. I 30 Paesi considerati nello studio sono stati classificati per macrogruppi, a seconda delle dinamiche registrate tra gli anni Ottanta e la prima decade del 2000. In questo quadro, l'Italia fa parte del gruppo dei Paesi mediterranei nei quali si evidenziano livelli di disuguaglianza abbastanza alti molto marcati. Lo studio considera, infine, gli effetti dei livelli di istruzione e delle dinamiche del mercato del lavoro sulla generazione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, che a sua volta incide sui comportamenti sociali e politici. La progressiva scolarizzazione nei Paesi sviluppati nell'arco dell'ultimo secolo ha ridotto le disuguaglianze nei livelli di istruzione, certo, ma questo non si è tradotto in un'effettiva riduzione anche delle disuguaglianze nei redditi, in quanto è mutato profondamente il mercato del lavoro. Si rileva, infatti, che i nuovi entrati nel mondo del lavoro sono certo più istruiti di un tempo, ma ora meno garantiti, quindi meno in grado di risparmiare e, pertanto, di assicurare redditi da capitale e da proprietà. È necessario perciò nel suo complesso ripensare una politica redistributiva ai fini della crescita e dello stesso sviluppo economico e un sistema distributivo che vada al di là degli interventi congiunturali, in quanto ci troviamo di fronte, come detto, ad una profonda crisi di sistema, che deve essere aggredita e affrontata con politiche strutturali e con un vero e proprio cambio di paradigma rispetto al più recente passato.

Da qui anche l'attesa per i prossimi possibili risultati dello stesso Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. Chiedo, infine, al primo firmatario della mozione n. 34 (testo 2) di poter aggiungere la mia firma.

Mi piacerebbe riportare il mio intervento a qualcosa già detto dal senatore Esposito nell'illustrare la nostra mozione, cioè a due parole fondamentali: la sussidiarietà e i tagli orizzontali.

sono gli enti più vicini ai cittadini che, secondo il citato principio di sussidiarietà orizzontale, erogano servizi ai cittadini. Questi servizi sono in continuo aumento e le risorse non bastano mai. Mi riferisco al sostegno educativo domiciliare per i minori, quindi ai nostri ragazzi, ai nostri figli,

degli anziani nelle case di riposo. Mi riferisco inoltre agli interventi economici finalizzati che i Comuni già erogano nei confronti dei cittadini al di sotto di un certo livello di reddito, naturalmente: anche in quel caso i Comuni non ce la fanno più con le risorse.

dati molto preoccupanti), e sappiamo che se non ci fosse il volontariato con la sussidiarietà orizzontale sarebbe impossibile dare risposte alle famiglie, provocando purtroppo quei fenomeni, che ci preoccupano, di tensioni sociali di cui si di cui si è qui parlato poc'anzi. Quindi, il concetto di sussidiarietà si unisce e va insieme a quello dei tagli orizzontali. Non è possibile più provocare tagli orizzontali nei bilanci perché quanto fa lo Stato poi viene fatto dalle Regioni, e poi dai Comuni, dai Comuni, in sequenza. Vorrei ricordare - non l'ho citato prima - anche il tema degli affitti e delle case che vanno alle famiglie con redditi bassi; anche qui tutti i fondi sono stati tagliati. Lo Stato, quindi, ha la necessità di intervenire in un doppio senso. evitare i tagli orizzontali, altrimenti gli enti locali si comportano di conseguenza. In presenza di tagli orizzontali, tutti i servizi di cui ho parlato prima (la domiciliarità per le famiglie e gli anziani,

gli anziani, che hanno costruito questo Paese, non ce la fanno i ragazzi a mettersi tutti sulla stessa linea nella corsa della vita. Questo è un concetto già richiamato, che noi non possiamo accettare. Senza la sussidiarietà e senza gli interventi menzionati naturalmente non si può proseguire. Poi serve un'inversione di tendenza, signora Vice Ministro: non si può procedere con l'assistenzialismo cronico.

Le persone che accedono agli interventi economici finalizzati devono avere l'obbligo, naturalmente sostenuti dai Comuni, di iscriversi ai centri per l'impiego delle Province, di

consideriamo davvero singolare la discussione di oggi contro la povertà. Non abbiamo ben chiaro se il tentativo dei soci di maggioranza del Governo è di prendere le distanze da quelle politiche di *austerity* che il Governo delle larghe intese sta portando avanti in piena continuità con i Governi Berlusconi e Monti, così come il senatore Monti ieri ha ricordato e precisato a tutti noi: scelte difficili e impopolari - ha detto Monti - che il Governo deve prendere per il bene del Paese. Ma quale sarebbe il bene del Paese? Le politiche di tagli e di *austerity* hanno finora solo prodotto impoverimento e rinviato la famosa crescita. L'Italia è un Paese ferito in profondità, è questa l'impietosa analisi del Rapporto sui diritti globali 2013 curato da forze sociali e del terzo settore: calano i consumi, le famiglie non riescono più a far fronte ai costi delle cure del medico e degli esami, non ce la fanno a pagare le bollette e il riscaldamento di casa. Cresce la povertà, mentre il rischio di esclusione riguarda ormai un quarto della popolazione. Tra il 2012 e i primi tre mesi del 2013 sono 121 le persone che si sono tolte la vita a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Oggi un terzo dei giovani non ha lavoro. Sono in atto oltre 160 crisi industriali, tra cui quelle dell'Ilva, della Lucchini e della FIAT. Il potere di acquisto è tornato ai valori di dieci anni fa e oltre 50 Comuni di media grandezza si trovano sull'orlo del dissesto finanziario. La povertà in Italia non è fatta solo di marginalità estrema, di cui parlava ieri il presidente Letta e di cui noi comunque ce ne facciamo carico, anche se non ha rappresentanza politica: oggi i poveri sono un'ampia fascia della popolazione, perché l'Italia in questi anni è diventato uno dei Paesi più diseguali d'Europa, con i salari medi diminuiti notevolmente. La disuguaglianza della società italiana si misura proprio nel divario crescente tra ricchi e poveri: ogni ricco ha il reddito di 100 poveri. Il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 45 per cento della ricchezza totale: una vera e propria piramide feudale che ha prodotto ingiustizia sociale e dunque disuguaglianza. Il peso del debito pubblico, l'obbligo all'austerità, i vincoli posti dall'Europa, la riduzione delle tasse, l'abbassamento delle tutele e dei diritti hanno prodotto una vittima sacrificale: il *welfare,* quello Stato sociale che negli anni passati ha segnato il passo delle politiche pubbliche di contrasto alla povertà. Ieri il presidente Letta ci ha detto che si esce dalla povertà con la centralità del lavoro; bene, affinché non risulti uno *slogan* sono necessarie politiche attive per il lavoro di qualità e dignitoso, lavoro per i tantissimi giovani disoccupati, le donne, gli inoccupati, per coloro che hanno perso il lavoro dopo i cinquanta anni e per la generazione dei trenta-quarantenni, quella generazione in ritardo: in ritardo per il lavoro e per la famiglia; in ritardo per la pensione, oltre che per i diritti, perché la precarietà è normalità. Occorrono scelte coraggiose e urgenti, a partire dall'eliminare la cosiddetta riforma Fornero che ha prodotto il disastro sociale degli esodati dei tanti mai pensionati della piccola e media impresa, riforma che non ha facilitato l'accesso ai giovani ai luoghi di lavoro, anzi, ha istituzionalizzato un grande conflitto intergenerazionale. Per consentire l'autonomia e la libertà di sottrarsi al ricatto della precarietà, soprattutto per i giovani, è necessario istituire finalmente il reddito minimo garantito: il diritto a quella esistenza libera e dignitosa prevista dall'articolo 36 della Costituzione. Si tratta di una misura prevista già in quasi tutti i Paesi d'Europa, con l'eccezione di Bulgaria, Grecia e Italia. Il reddito minimo è riconosciuto a tutti come un diritto soggettivo; ne beneficiano coloro che non hanno un lavoro o hanno un reddito basso, come avviene in Paesi come la Germania. Diciamo di voler raggiungere gli *standard* europei, ma non siamo consapevoli di rappresentare un'eccezione in Europa: disoccupazione e precarietà non significano la stessa cosa in Francia,

Combattere la povertà vuol dire fondi per l'infanzia, l'immigrazione e la famiglia; fondi, ad esempio, per l'agricoltura sociale, per promuovere le attività agricole, per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio, per promuovere lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali, contrastando così la politica dei tagli ai servizi sociali e cogliendo le grandi opportunità che offre l'agricoltura multifunzionale. Contrastare la povertà deve voler dire rifinanziare il Fondo per la non autosufficienza. Averlo azzerato è stata un atto di barbarie, crudeltà ed emarginazione.

e si capisce come mai aumentino coloro che rinunciano alle cure e ai farmaci a causa del loro costo. Fermare l'aumento indiscriminato dei *ticket* e allargare i LEA, inserendo le cure odontoiatriche: sono in aumento coloro che rinunciano a curare i denti per gli elevati costi cui non è possibile più far far fronte (e tra questi molti bambini). Sono in aumento le persone che subiscono uno sfratto. Siamo un Paese che investe in diritto alla casa lo 0,1 della spesa sociale e in dieci anni abbiamo tagliato il 95 per cento del fondo che sostiene l'affitto. Non siamo in grado di garantire alcunché anche a persone che lavorano e hanno un reddito, ma non ce la fanno. Così dei 290.000 sfratti emessi negli ultimi cinque anni, ben 240.000 sono per morosità e molti altri ancora ne vedremo nei prossimi anni. È urgente dunque un piano di edilizia sociale pubblica di qualità, utilizzando l'esperienza dell'autocostruzione, recuperando edilizia da rottamare e dando alloggi ad affitto sociale. Naturalmente è necessario liberare gli enti locali dai vincoli del Patto di stabilità e il nostro Paese dalla morsa anticostituzionale del *fiscal compact*. Noi, a differenza di quanto è stato detto ieri in questa Aula, saremmo molto contenti se il presidente Letta riuscisse ad aprire in Europa un varco su questi temi: vorrebbe dire restituire risorse alle Regioni e agli enti locali per politiche vere di contrasto alla povertà, politiche di inclusione e di buona cittadinanza, politiche che possono e devono vedere il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali, del ricco mondo del terzo settore, ma in un rapporto di sussidiarietà chiara, che non deve scadere in corporativismo e consociativismo, attraverso progetti di accoglienza, inclusione e integrazione, e non per la distribuzione delle *card*. Riforme strutturali, dunque, e non interventi caritatevoli, che rischiano un'ennesima parcellizzazione delle risorse. Soltanto dando centralità vera al lavoro, usando la leva fiscale per ridistribuire la ricchezza, come previsto dall'articolo 53 della Costituzione, superando il *fiscal compact*, investendo in sanità e politiche sociali, introducendo il reddito minimo garantito,

le politiche sociali adottate negli ultimi anni dal nostro Paese risentono della mancanza di un elemento fondamentale, quello della prospettiva. La mancanza di tale comun denominatore si ritorce contro chi dovrebbe essere l'oggetto attivo di tale intervento, ovvero i giovani. Secondo gli ultimi dati ISTAT citati dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel rapporto annuale presentato il 10 giugno scorso, in Italia vivono in situazione di povertà relativa ben 1.822.000 minorenni, per cento dei bambini e degli adolescenti, e il 7 per cento dei minorenni vive in condizione di povertà assoluta. Preoccupante è anche il rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni, pari al 70 per cento nel Mezzogiorno. Inoltre, come la ministra Carrozza ha detto, la mancanza di mezzi non può continuare a tradursi sempre di più in esclusione sociale e culturale, e la dispersione scolastica e la disoccupazione sociale sono intimamente collegate. poi anche il minor ricorso alle cure sanitarie a preoccuparci tantissimo; questo mette a rischio un aspetto importantissimo nel nostro Paese, in cui si sono compiuti davvero passi da gigante, quello della prevenzione. Costituisce dunque un grande rischio la povertà. Come affermato dal Garante, la crisi economica e sociale che negli ultimi anni l'Italia e il resto del mondo stanno affrontando non può essere l'unica causa di

ha poi avuto una ricaduta anche nei Comuni che devono garantire i servizi, non ha fatto altro che peggiorare tale situazione. Come sostenuto giustamente dal presidente Grasso, noi siamo di fronte ad un impoverimento morale, dove le parole giustizia, cultura e tutela dei diritti fondamentali sembrano essere scomparse dal vocabolario e dal tessuto sociale. Seppure il progresso e l'impegno, già citato, da parte del terzo settore e del volontariato sociale hanno permesso il raggiungimento di alcuni importanti traguardi in questo campo, moltissimo resta ancora da fare.

questa ottica un primo passo per la lotta alla povertà minorile, a partire dalle famiglie più marginali, rispetto al mercato del lavoro. La sperimentazione di questa nuova *social card*, avviata dal decreto interministeriale del 10 gennaio 2013, consiste in un trasferimento monetario riservato a famiglie in condizioni di povertà residenti nei 12 Comuni con più di 250.000 abitanti. Vede, collega Catalfo, ritengo che comunque la

si misura l'efficacia del programma confrontando i risultati raggiunti dal gruppo dei soggetti beneficiari rispetto alla situazione del gruppo, statisticamente confrontabile, che però non ha partecipato a questa sperimentazione. Durerà un anno e la gestione sarà infine affidata ai Comuni. Il Governo ha stanziato un *budget* di 50 milioni di euro che saranno ripartiti tra i Comuni in base all'incidenza della povertà assoluta rilevata dall'ISTAT nelle diverse aree del Paese. Tale programma è rivolto a famiglie in difficoltà. Rispetto alla vecchia carta acquisti ci sono dei vantaggi: la vecchia carta acquisti era riservata alle famiglie con anziani e a quelle con bambini di età inferiore ai tre anni

un abbattimento, contro l'assistenzialismo diffuso e cronico. Alcuni aspetti sono indubbiamente migliorabili; indubbiamente, mi sento di dire alcune cose. La prima suggestione è che la povertà può essere causa di pericolose tensioni sociali. La seconda, signor Presidente, è che la scarsa partecipazione alla vita democratica di intere fasce di popolazione, escluse a causa della dispersione scolastica che non permette l'accesso ad ad un livello culturale degno, delegherà di fatto a pochi il compito di rappresentanza. Concludo il mio intervento citando, di nuovo, il presidente Grasso, oggi fonte per me di Per risolvere quella che il presidente Grasso definisce una vera è propria questione sociale dobbiamo porre, anche attraverso questa mozione

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutto ci saremmo aspettati tranne che nel nostro Paese ci si dovesse trovare in Parlamento ad affrontare una mozione con la quale impegnare il Governo ad adottare misure urgenti finalizzate ad arginare la crescita esponenziale del fenomeno della povertà. Ingenuamente pensavamo che la povertà dovesse essere classificata come una condizione estrema dovuta a fattori esterni ben identificabili e relegata soltanto a determinate categorie e classi sociali svantaggiate. La crisi economica internazionale che si è abbattuta violentemente anche sul nostro Paese ci ha aperto gli occhi e ci ha consegnato uno scenario di forte depressione e recessione che ha causato una lenta ed inesorabile diffusione della povertà. Le misure correttive per risanare i conti messe in atto dai Governi che si sono succeduti dal 2007 (anno di riferimento dell'inizio della crisi ad oggi) hanno prodotto un precario equilibrio nei bilanci di quei cittadini e quelle famiglie dapprima considerati classe media, esponendoli al rischio povertà. Tra le misure correttive ricordiamo: la crescita dell'imposizione fiscale, che - va ricordato - è andata ad incidere anche su un bene primario come la prima casa;

termine osceno frutto della fantasia dei commentatori della politica, ma dietro il quale si celano situazioni di enorme sofferenza. Parliamo di persone con un nome e un cognome, dei figli e dei nipoti che, da un momento all'altro, si sono ritrovate senza alcun reddito e che, nei casi peggiori in cui non vi era la possibilità di far ricorso ai risparmi, sono state catapultate in una condizione di indigenza. questo vanno aggiunti logicamente i tagli alle risorse operati agli enti locali che hanno inevitabilmente inciso sull'efficienza delle strutture e sugli interventi mirati ai servizi alla persona. le crisi economiche sono cicliche, come del resto tutti gli eventi drammatici che caratterizzano la storia di un Paese. Se ciò è vero, è altrettanto vero che questa crisi era stata ampiamente preannunciata. Era dinnanzi agli occhi di tutti che le politiche economiche che hanno caratterizzato gli anni Novanta, diciamo dal crollo del Muro di Berlino ad oggi, fossero improntate sul nulla! Una finanza creativa fondata sul niente, un castello costruito sulla sabbia. Un'errata presunzione, fondata su un processo logico-alchemico (quello che con i soldi si potessero fare altri soldi), accompagnata dall'incapacità politica di imporre delle regole ai mercati e dei limiti all'attività della grande finanza, fondata principalmente su modalità speculative, ha prodotto inesorabilmente il disastro che stiamo vivendo. La cosa ben più grave è che da tutto ciò poco si è imparato. Gli interventi politici messi in atto al fine di contrastare questa crisi si sono incentrati principalmente su aiuti strutturali o meno verso le banche d'affari e i grandi istituti finanziari e per di più per far ciò si sono messe in atto misure di contenimento dei costi, che hanno avuto forti ripercussioni proprio sui cittadini e le famiglie facendo diminuire il loro potere d'acquisto. Coloro che hanno causato la crisi sono stati premiati e questo premio è stato materialmente costruito sulla pelle dei cittadini. Tutto ciò è incredibile; tutto ciò è assurdo, come è assurdo che per quasi due anni le sorti del nostro Paese siano state letteralmente commissariate: le decisioni politiche del Governo Monti - va ricordato - erano assoggettate alle decisioni prese dai burocrati europei. Era un Governo - come più volte detto - non scelto dal popolo e che rappresentava soltanto ed unicamente gli interessi dei poteri forti; un Governo che con le sue scelte scellerate ha contribuito unicamente al peggioramento della situazione, come facilmente dimostrabile dall'analisi dei principali fattori macroeconomici; un Governo che, come Lega Nord, abbiamo contrastato fin dal primo giorno del suo insediamento, con senso di responsabilità e non venendo mai meno alla parola data ai nostri elettori. Critici e convintamente all'opposizione, siamo consci che lo scenario attuale, pur non essendo quello auspicabile, è comunque differente. Questo Esecutivo, difatti, a noi non piace e siamo certi del suo inevitabile fallimento, ma, a differenza del precedente, non possiamo non constatare che questo è un Governo politico; per questa ragione con la nostra mozione lo vogliamo impegnare a prendere posizioni politiche. Avviandomi alla conclusione, lasciate che in quest'Aula - come più volte precedentemente ricordato vi dica chi sono, da dove vengo, dove affondano le mie radici, cosa mi abbia spinto ad entrare in politica e ad essere parte attiva di questa rivoluzione del sistema, in un'ottica federale che incarna il movimento della Lega Nord, di cui mi onoro di far parte. È ben noto a tutti che prima di sedere sugli scranni del Parlamento ero un'operaia. Sì, sono onorata ogni volta si presenti l'occasione di ricordare che io sono stata e sono un'operaia. "sono" e "sono stata" perché poco è cambiato. Prima mi sentivo partecipe di un processo nel quale con il mio lavoro contribuivo a portare alla luce un prodotto da immettere sul mercato; l'uomo nasce, infatti, consapevole che proprio grazie al suo ingegno e al suo sudore può creare e costruire ciò di cui ha bisogno per la sua sopravvivenza; oggi sono un'operaia del mio movimento ed il mio operare è incentrato sulla necessità di offrire un contributo per la ricerca del bene comune. Ho sentito la necessità di parlare della mia personale esperienza proprio per rendere palese come mai e poi mai si potrà assicurare una tranquilla esistenza alle generazioni future fino a quando la politica non si riapproprierà del suo ruolo e si scrollerà definitivamente quella soggezione che la rende succube degli interessi esercitati dai cosiddetti poteri forti. Sono a sottolineare come sia corretto e doveroso impegnare il Governo ad operare interventi urgenti, finalizzati a prevedere misure di contrasto alla povertà anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse economiche da destinare in particolar modo al territorio, essendo difatti proprio le Regioni e gli enti locali i primi soggetti chiamati ad intervenire in quelle politiche di *welfare* che si concretizzano in aiuti alla popolazione, piani di contrasto all'emergenza abitativa, aiuti diretti alle famiglie (in particolar modo, a quelle numerose), ai portatori di *handicap*, ai genitori separati, insomma a tutte quelle fasce di popolazione particolarmente deboli. Detto ciò, penso sia veramente vitale ribadire in questa occasione, attraverso la formulazione esplicita di un impegno, l'esigenza che il Governo si faccia promotore, in tutte le sedi competenti, di una rinnovata linea politico-programmatica fondata sulla necessità di operare un vero e proprio cambiamento dell'attuale sistema.

cioè ridare quella differenza tra il potere reale e commerciale della moneta al popolo italiano. Basterebbe quindi non fare grandi discussioni, ma prendere una proposta di legge che è già stata presentata, portarla in discussione nelle Commissioni, votarla e restituire a quella Banca d'Italia, che una volta era degli italiani, aiutava i figli dei lavoratori, dava la possibilità di costruire case popolari e consentiva alle piccole e medie imprese di poter operare, la possibilità a una situazione di normalità. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, basterebbe restituire la Banca d'Italia agli italiani e togliere ai banchieri quella quella differenza tra potere reale e potere commerciale della moneta, che su 500 euro è pari a 499,80 euro. Basterebbero piccole cose per ridare ossigeno all'Italia, far ripartire l'economia di questo Paese e dare risposte serie nell'interesse

È iscritta a parlare la senatrice D'Adda. Ne ha facoltà. tra i tanti dati economici che purtroppo possono essere evidenziati nel difficile presente che il nostro Paese sta vivendo, ce n'è uno che viene troppo spesso sottovalutato, ma che invece dovrebbe essere il primo a il primo a spingerci a riflettere sulla gravità della situazione odierna e a promuovere interventi immediati e decisivi. Mi riferisco alla diminuzione drammatica dei consumi alimentari, tendenza negativa che dura ormai da cinque anni

Basterà comunque ricordare il rapporto diffuso nell'ottobre 2012 dalla Caritas per fugare ogni dubbio al riguardo. La Caritas evidenzia infatti come tra le persone che si sono rivolte ai suoi centri nel 2011 vi sia un aumento significativo tra categorie che sino che sino a poco tempo fa non erano interessate in misura così pregnante dal rischio povertà: sempre più italiani, sempre più ex ceto medio. Per avere ulteriori prove di ciò che sta succedendo ci si potrebbe soffermare nel nostro quotidiano, o almeno in quello di chi va a fare la spesa.

possibilità economiche perché, per intendersi, i soldi sono finiti. Si tratta di una crisi economica che, come più volte sostenuto, si aggrava proprio a seguito del crollo di quella propensione al consumo nel mercato interno, a sua volta fortemente condizionata dall'incertezza e dalla precarietà del mercato del lavoro. L'incertezza e la paura del futuro fanno contrarre la propensione al consumo, con effetti drammatici sull'economia reale e l'occupazione. Il lavoro diminuisce e quando c'è risulta spesso sottopagato. La pressione fiscale aumenta per mantenere fede agli accordi europei e la povertà inevitabilmente cresce e interessa sempre più anche il ceto medio. il lavoratore post-fordista, come, tramite un eufemismo, potremmo chiamare il lavoratore flessibile e precario (quello che ci ritroviamo oggi da tutte le parti), si trova di fronte alle esigenze della propria esistenza privo della pur minima protezione sociale; ciò comporta forti squilibri, soprattutto nella gestione della propria vita presente e nelle scelte per il futuro. La psicologia della scarsità, che da questa situazione di crisi e precarietà deriva, genera ansia, invidia, egoismi e disagio sociale. Ecco allora che anche in Italia, come già succede diffusamente in Europa, è urgente e necessaria l'introduzione del reddito minimo garantito. Non fosse altro, un po' cinicamente, per gli effetti benefici che una tale misura avrebbe immediatamente dal punto di vista dei consumi interni. È risaputo infatti che la propensione al consumo è elevata quando a beneficiare di incrementi di reddito sono persone con difficoltà economiche, in quanto sono maggiori i bisogni primari da soddisfare. D'altra parte, è d'obbligo far notare come non si veda quale migliore misura potrebbe essere adottata dall'Italia per raggiungere gli obiettivi che si è posta.

Si dirà a questo punto che mancano i soldi e che i vincoli europei ci impediscono di intervenire in questa direzione. In realtà, tutto dipende da come si decide di intervenire, e i costi non devono diventare l'ennesimo alibi affinché nulla cambi, la solita teoria del Gattopardo, che conosciamo più o meno tutti per cui tutto cambia perché nulla cambi. Proprio dal lato dei costi, ad esempio, è interessante la relazione del 2011 sui risultati e sui costi del

1,8 milioni di famiglie, circa 4 milioni di individui, di cui il 64 per cento risultava del tutto privo di reddito, mentre il 36 per cento ha richiesto il sussidio integrativo. La spesa complessiva per il finanziamento del *revenu de solidarité active* in Francia, nel 2010, è stata di 9,8 miliardi di euro. È una cifra molto simile a quella che l'erario italiano spende attualmente per i suoi ammortizzatori sociali. Secondo la UIL, infatti, nel 2011 le indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione sono costate nel complesso 18 miliardi di euro, di cui ben 9 miliardi hanno pesato sulla fiscalità generale. significa che abbiamo speso, per un sistema di *welfare* che tutela solo un lavoratore su due, la stessa cifra che in Francia ha garantito a tutti un programma di protezione universalistico e più equo. Del resto i vincoli europei alla spesa non possono essere utilizzati come alibi anche per un altro motivo. Sono state proprio le istituzioni della Comunità europea,

Dalla prossima volta richiamerò i colleghi nominalmente, in modo che a casa si sappia che il collega è presente, ma anche che cosa sta facendo. *(Applausi dal ringrazio, signor Presidente. Non sono una grande oratrice: questo è un Parlamento e dobbiamo parlare, però qualche volta proviamo ad ascoltarci un poco. Del resto i vincoli europei alla spesa non possono essere utilizzati come alibi anche per un altro motivo. Sono state proprio le istituzioni della Comunità europea, infatti, a indicare in più occasioni agli Stati membri la necessità di introdurre programmi nazionali di lotta alla povertà e all'esclusione sociale che prevedessero strumenti universalistici

che ne salvaguardi la dignità sociale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede all'articolo 34, terzo comma, il diritto di ognuno (cittadino europeo o residente stabile nel territorio dell'Unione) all'assistenza sociale e abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. In attuazione della Carta di Nizza, il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»; la mancanza di garanzie e di diritti non solo genera un nuovo disagio sociale e nuove povertà, ma rimette in discussione quel piano di riconoscimento della cittadinanza, di appartenenza ad una comunità democratica. Ecco perché il reddito minimo garantito deve essere riconosciuto come un diritto del cittadino, inserito in un contesto più ampio di nuovi diritti-doveri e nella costruzione di un nuovo immaginario di società. Senza un reddito minimo garantito, con le enormi disparità economiche presenti oggi, con la forte polarizzazione dei redditi e l'enorme precarizzazione, rischiamo di avere una democrazia a metà, un sistema che vede le disparità sociali riemergere con forza. L'Europa che a noi piace è l'Europa che riconosce questi diritti e agisce di conseguenza con misure di sostegno al reddito; un'Europa in cui l'Italia non è ancora entrata, nonostante abbia dato i natali a due persone che già nel 1941 scrivevano queste parole: «La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica, non dovrà manifestarsi con le forme caritative sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro vessatori». Coloro che hanno pronunciato queste parole erano Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e, nella loro idea di Europa, come nella nostra, almeno del nostro Movimento, nessuno deve rimanere indietro.

nel momento storico che ci troviamo a vivere, di profonda crisi e incertezza per numerose famiglie e lavoratori del nostro Paese, è essenziale e prioritario dare una risposta forte da parte nostra per contrastare la povertà che colpisce nuove categorie e classi sociali, senza distinzioni. Occorre, però, dare risposte innovative e concrete alla questione, ed affrontare il problema non solo in termini finanziari ma anche e soprattutto culturali. Insieme alle nuove povertà, infatti, stanno emergendo nuovi fattori di rischio sociale: l'isolamento, il degrado e la paura. la Caritas, nel suo rapporto annuale, ha evidenziato che sempre di più i nuovi poveri sono categorie considerate fino a qualche anno fa come classe media che riusciva ad arrivare a "fine mese" dignitosamente.

Siamo però anche consapevoli che questo è un momento estremamente difficile per il bilancio dello Stato, nell'ambito del quale non si riesce a reperire nuove risorse per affrontare le sfide che la crisi ci chiede di affrontare. Noi siamo contro i tagli lineari, che colpiscono anche e soprattutto questa spesa necessaria e vitale, cioè quella sociale, e quindi c'è più che mai bisogno di un atteggiamento responsabile, che consenta non solo di tagliare la parte di spesa pubblica improduttiva ma anche di responsabilizzare i centri erogativi. Lo Stato si trova nella condizione di non potersi permettere di fare tutto quello che faceva prima; bisogna perciò sfruttare al meglio le risorse e le possibilità che abbiamo a disposizione. Quindi, bisogna aiutare e sostenere chi già lavora e conosce bene la situazione delle famiglie italiane colpite dalla crisi; bisogna valorizzare tutte quelle esperienze positive già sperimentate ed attive sui territori, riconoscendo il ruolo dei corpi intermedi, che svolgono un'importante azione a sostegno delle fasce più deboli della società e sono direttamente a contatto con le situazioni drammatiche che larghi settori della nostra società vivono quotidianamente. Come ci ricordava infatti Madre Teresa di Calcutta, «Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i poveri». E noi proprio coloro che parlano con i poveri dobbiamo valorizzare, perché bisogna partire dal presupposto che essere poveri oggi non significa ovunque la stessa cosa. Pertanto, la conoscenza profonda ed accurata di ogni singolo contesto locale e la vicinanza alle persone che in quel contesto vivono e soffrono sono i prerequisiti necessari di qualsiasi programmazione o intervento contro la povertà; caratteristica, questa, propria dei nostri servizi sociali e soprattutto del mondo del volontariato, settori che oggi si trovano in profonda difficoltà nel far fronte alle continue e nuove richieste di aiuto. È prioritario, quindi, applicando il principio della sussidiarietà, aiutare e sostenere i nostri enti locali, il mondo dell'associazionismo e del *non profit*, agendo a loro sostegno sia dal punto di vista legislativo che fiscale e agevolando il loro lavoro nell'aiuto quotidiano a sostegno dei cittadini dei cittadini italiani, perché arrivano dove lo Stato non riesce o non può arrivare. Quindi, dicevamo, riconoscere e valorizzare questo aspetto positivo ed operoso della nostra società. Ma a tutto ciò devono essere accompagnate scelte economiche e politiche sane ed efficaci, che non trascurino la natura della persona né la sua dignità e siano orientate alla giustizia sociale e alla solidarietà.

In questo senso, nulla ha a che vedere con l'assistenzialismo cronico, che tutti noi siamo convinti debba essere combattuto per liberare risorse. La morosità incolpevole è frutto di una crisi veramente devastante

da Sud verso Nord. Quindi, anche le Regioni più ricche soffrono, sia pure in percentuale minore, questo problema. Vengono attuati sfratti anche dagli istituti di edilizia residenziale. Da questo punto di vista sappiamo che nemmeno i Comuni possono più intervenire, perché chi è sfrattato da un istituto delle cosiddette case popolari non può più fare domanda, addirittura, se non dopo cinque anni. Abbiamo necessità di fare due cose: i fondi attualmente stanziati sono troppo esigui,

che qui sono stati ricordati - e che non voglio ripetere, altrimenti porterei via tempo - è, però, indispensabile intervenire anche con alcune misure che possano essere spendibili subito sul territorio. In questo senso, abbiamo bisogno che, insieme a noi, dialoghino anche i sindacati, l'ANCI, in rappresentanza di tutti i Comuni, e, anche la Conferenza delle Regioni, altrimenti da questa situazione non riusciremo ad uscire. Ribadisco in questa sede un dato che mi pare davvero fondamentale: l'uscita dalla crisi e la lotta alla povertà possono avvenire soltanto se noi tocchiamo, punto per punto, il rivolgimento della struttura fiscale e di intervento della nostra comunità. Se non facciamo questo, non riusciremo a uscirne. Se non interveniamo da subito con alcune misure tampone, sono del parere che non riusciremo ad aiutare gli enti locali, che in questo momento non trovano risposta neppure alle questioni, come il *social housing*, che aggrediscono solamente in minima parte il problema. allora, i punti più importanti, non lasciamoci fuorviare dall'ideologia e diamo una risposta positiva alle mozioni che, da subito, vogliono dare respiro a chi in questo momento non ha più nemmeno la possibilità di guardare un tetto, ma guarda soltanto un cielo aperto.

Il sentimento che è stato espresso è fondamentalmente comune, così come comune è la convinzione che il contrasto alla povertà debba coinvolgere l'intera filiera istituzionale, dal Governo centrale, alle Regioni e ai Comuni, come enti di vicinanza, e tutto il terzo settore. Ciascun Gruppo ha ovviamente fatto le proprie sottolineature e ha dato anche indicazioni sulle diverse formule

vedere se il Parlamento riesce a trovare un'unità nell'esprimersi su questo tema così delicato ed importante. Un elemento comune è che si debba assumere, sia pure nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e con un passaggio

Colgo l'occasione per dare un'informazione su un tema che ricorre in varie mozioni presentate e che riguarda la distribuzione del fondo nazionale delle politiche sociali.

in generale, che le norme che non riguardano specificamente la questione sociale siano espunte dalle mozioni. In particolare, per quanto riguarda questo profilo - che si ritrova anche in un'altra mozione - ricordo che nella delega fiscale, che sta riprendendo il suo cammino in Parlamento, un punto

fortemente decrescente, per cui non è plausibile ritenere che, da un aumento delle aliquote, si abbia un aumento di gettito. In questa situazione, e per le caratteristiche di quel tipo di prelievo, probabilmente si avrebbe, al contrario, una diminuzione.

avviare, in tempi rapidi, tutti i necessari interventi per rendere attuativo il federalismo fiscalecosì da garantire anche interventi destinati a migliorare le condizioni delle fasce deboli della popolazione, in primo luogo le famiglie

nell'ottica di non vincolare in modo troppo stretto le politiche che si stanno intraprendendo, salvaguardando però tutte ispirazioni di cui abbiamo parlato prima,

non determinare un'intera finalizzazione comune del finanziamento sociale e di quello sanitario, dal momento che hanno specificità che si ritiene debbano essere salvaguardate, ma sicuramente prevedendo anche fonti di finanziamento integrato. di riformulare il punto 4) del dispositivo in questo senso: «ad utilizzare la carta acquisti come strumento nel contrasto alla povertà e l'esclusione sociale, coinvolgendo nella strategia di contrasto anche gli enti locali e le organizzazioni non profittevoli».

che sollevo lo porrò anche con riferimento all'ordine del giorno, ed è quello di non vincolare il Governo a una specifica dizione, che sappiamo essere divisiva, ma di impegnarlo con forza a introdurre, per quanto per gradi, misure di contrasto alla povertà assoluta.

individuando categorie specifiche di intervento, propongo di espungerlo e di trattare tale argomento nel contesto delle politiche attive del lavoro. Tra l'altro, come sapete oggi il Governo assumerà misure esattamente su questo tema, che saranno quindi oggetto di confronto e di dibattito in Parlamento,

con la massima urgenza e con decisione, un percorso che porti all'introduzione progressiva nel nostro Paese di una misura strutturale di contrasto alla povertà», riprendendo in tal modo un elemento che è stato sottolineato in diversi interventi, cioè il fatto che uno dei limiti dell'intervento di contrasto alla povertà nel nostro Paese è proprio la mancanza

alla fine un lungo elenco, più o meno condivisibile, di misure strutturali che dovrebbero essere messe in campo per contrastare la povertà, ma viene meno la particolarità

come la *social card*, le cui sperimentazioni (fatte precedentemente sotto altri nomi) non sono un ricordo a cui richiamarci nella storia recente di questo Paese, senza nulla togliere a quel grande momento di umiliazione sociale da queste esperienze. Noi ovviamente riteniamo più giusto operare perché si realizzino nuovi modelli di sviluppo dove i cardini fondamentali siano eguaglianza e giustizia.

Signor Presidente, signora Vice Ministro, onorevoli colleghi, in un'Europa colpita dalla grave crisi economica e finanziaria, è doveroso che chiunque voglia mettere a disposizione tempo ed energie al servizio del popolo nell'attività politica tragga ispirazione dalla difesa dei valori identitari e si impegni per la tutela di quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e beni che rappresentano il motore di un Paese civile. doveroso ricordare come l'attuale crisi economica abbia origine dal crollo dei mutui *subprime* dell'estate 2007 con il conseguente fallimento a catena di alcune banche di affari che, senza alcuna regolamentazione e per giunta con la copertura ufficiale delle agenzie private di certificazione, operavano attraverso fraudolenti meccanismi di speculazione finanziaria. Tra le cause principali dell'attuale crisi vi è il fallimento di un modello economico e politico, nel quale le istituzioni hanno abdicato il loro ruolo di garanti delle regole al potere esercitato dalla finanza e dalla grande industria. un cancro diffuso in tutti i settori, che vede però il concentrarsi delle sue metastasi proprio in quelle operazioni speculative messe in atto dalle agenzie di intermediazione finanziaria. La così tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è dimostrata totalmente fallimentare. Il sistema finanziario e monetario, sempre più deregolamentato e sottratto ai controlli preposti, ha minato ogni forma di *governance*, dando così origine ad una serie di bolle finanziarie distruggendo i settori industriali, commerciali e agricoli produttivi. Questo scenario di crisi è stato, inoltre, accompagnato da una evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi, inclini alla corruzione e alla collusione, alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica. Si è generato così in molti cittadini - troppi direi - un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori. Tutto ciò preoccupa. Sono e siamo convinti, infatti, che non vi sia altra strada per uscire da questa crisi economica e valoriale, se non quella di restituire alla politica il suo ruolo centrale: una politica intesa come spazio pubblico in cui si manifesta l'azione umana, imprescindibile dall'etica. Assistiamo, al contrario a una delegittimazione della politica. La politica è male e, in quanto tale, deve essere debellata. Il pensiero dell'antipolitica che si sta diffondendo velocemente, alimentato ad arte da una comunicazione scorretta che ha venduto la sua onestà intellettuale al potere di turno, dalla strategia del terrore diffusa dai tecnici al servizio della grande finanza e dalla irresponsabile gestione della cosa comune affidata a politicanti da circo, sta producendo danni irreparabili. Stando, infatti, ai dati elaborati e pubblicati dai principali istituti scientifici, dalle associazioni di categoria e dei consumatori, nel nostro Paese diminuiscono in modo drastico i consumi, anche quelli riferiti ai beni alimentari, come è stato evidenziato, mentre aumenta in modo esponenziale il numero dei disoccupati, degli inoccupati e dei cassaintegrati,

Per dare una risposta a tutto ciò è ovvio che sia necessario promuovere nel breve periodo interventi straordinari, diretti ad incrementare le risorse da destinare alle politiche mirate a contrastare la diffusione della condizione di povertà vissuta da molti cittadini e famiglie. che si prevedano misure di sostegno alle politiche economiche degli enti locali, che hanno la responsabilità diretta di quel *welfare* territoriale che si presenta come prima, reale e concreta struttura per sviluppare una rete di aiuti concreti alla popolazione. La recente esperienza deludente del progetto di Costituzione dell'Europa unita dovrebbe servire da monito per dare come assiomatico il presupposto che la politica non può essere sostituita. È oramai evidente il miserabile fallimento di dar vita ad una Europa unita, oggi fondata esclusivamente su criteri economicistici. Un'Europa che si è dotata di una moneta unica ancor prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica e sociale. Un mostro che, come nel mito di Kronos, si è nutrito dei suoi stessi figli. Questa Europa, plasmata in modo ideologico dal potere della grande finanza e privata di qualsiasi riferimento storico e culturale, ha generato, infatti, un diffuso sentimento critico nei suoi stessi confronti, tanto che, ogni qualvolta è stato possibile sottoporre a *referendum* la ratifica di un trattato comunitario, l'esito è stato puntualmente negativo. Ma per far tutto ciò è necessario con coraggio ammettere il fallimento dell'attuale sistema ed adoperarsi in tempi rapidi per fornire a questo Paese una via d'uscita. È necessario, infatti, che si provveda immediatamente a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all'applicazione di quanto definito nella riforma sul federalismo fiscale.

Questa riforma interviene sull'assetto dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti locali, modificando in profondità il modello che ha regolato, fino ad ora, il finanziamento degli enti territoriali, al fine di rendere migliore il funzionamento delle amministrazioni, la qualità della spesa e gli equilibri di finanza pubblica. Un sistema innovativo, nel quale, superati i trasferimenti, le risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo per i territori a minore capacità fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 prevede il passaggio graduale dal finanziamento basato sul criterio della «spesa storica» a quello, necessario e fondamentale, determinato in relazione al cosiddetto fabbisogno *standard*. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* è finalizzato, in ultima istanza, ad orientare la politica delle amministrazioni comunali verso una nuova logica meritocratica, che eviti le note inefficienze del passato e introduca nuove logiche manageriali di gestione delle risorse pubbliche. È una rivoluzione culturale che richiederà, anche da parte delle amministrazioni comunali, un notevole sforzo di cambiamento delle tradizionali formule amministrative, ma che sicuramente nel medio-lungo periodo determinerà un miglioramento complessivo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi destinati alla persona. È evidente come, attraverso questo approccio, si possa promuovere un cambiamento radicale del governo locale e, quindi, dell'intero Paese. Un percorso articolato e progressivo che verrà completato con l'approvazione di una complessiva riforma che ridefinisca le funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di semplificare, ridurre i costi e consentire un maggior controllo da parte dei cittadini, stabilendo, attraverso la definizione dei criteri di sussidiarietà orizzontale e verticale, le modalità con le quali lo Stato può trasferire le ulteriori funzioni amministrative. Una riforma che inevitabilmente comporterà consistenti risparmi di spesa per la macchina pubblica e un complessivo snellimento delle strutture amministrative e che permetterà ai cittadini di sentirsi realmente vicini ai propri amministratori. Questa nuova autonomia regionale e locale sarà guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi, quello del *favor familiae*: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti». Si tratta di principi altamente innovativi che connotano questa riforma nella direzione di un maggiore riconoscimento dei carichi familiari e quindi nella direzione di una maggiore attuazione del *favor familiae* che orienta il nostro dettato costituzionale. Per dare un segno decisivo di cambiamento bisogna innanzi tutto che la società si riappropri di quei principi e valori insiti nella tradizione religiosa, etica e culturale del nostro Paese. Riappropriarsi di questi valori fondanti della nostra società significa in primo luogo riaffermare la forza insita nell'istituzione della famiglia. Per noi è irrinunciabile l'esigenza di difendere la famiglia non a parole, ma con atti e scelte politiche chiare. È doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico, attuare le condizioni necessarie affinché nell'ambito della stessa famiglia possa realizzarsi la compresenza di più generazioni, favorendo la permanenza delle persone anziane nel nucleo familiare. La tutela dell'istituzione famiglia e la valorizzazione della missione politica sono gli assiomi dai quali partire per rifondare quel sentimento identitario e culturale del nostro popolo e dar vita finalmente ad una rinnovata Unione europea: l'Europa dei popoli. *(Applausi dal

ci ha dato la possibilità di confrontarci su tematiche estremamente scottanti, che coinvolgono la realtà sociale non solo italiana, dove fragilità e vulnerabilità rientrano nel diario della quotidianità. Più che dare una declinazione, in un vocabolario di terapie, in termini di contrasto alla povertà, è a me molto più caro in questo momento richiamare i fondamenti, i principi di riferimento che possono rappresentare a noi tutti la bussola con la quale affrontare i marosi di una crisi estremamente pervadente e invadente, che rende possibile, anche per realtà sociali che fino a qualche mese or sono potevano godere di uno stato di parziale benessere, di trovarsi in situazione di notevole disagio. Se dovessimo chiederci qual è il fondamento del vivere sociale, diremmo che sicuramente è quello della dignità della persona umana. da un lato, il fondamento del sociale e quindi del politico ma, dall'altro, rappresenta anche l'obiettivo che noi dobbiamo perseguire. Non dobbiamo andare molto lontano per riguadagnare quella strada che ci è stata tracciata da tempo, i cui principi e valori di riferimento da parte nostra possono essere coniugati nella quotidianità, ma anche nello sviluppo dell'azione politica. Queste parole sono socialità e sussidiarietà, libertà e responsabilità. Su di una in particolare mi vorrei soffermare, perché ritengo che il tema della sussidiarietà rappresenti il fondamento, il *leitmotiv*, il filo conduttore non solo degli interventi che mi hanno preceduto, ma sicuramente di quello che rappresenta il DNA di Scelta Civica per l'Italia. Qual è la legge fondamentale del principio di sussidiarietà? Ha un grande valore di eticità, nel senso che ciascuno è se stesso attraverso l'altro, attraverso il conseguimento del benessere dell'altro, del benessere nel senso psicofisico, sociale ed economico. Questo sta a intendere anche che il benessere dell'altro diventa benessere mio personale.

Si è così declinata la vita politica su queste tematiche, nell'ambito del contrasto alla povertà, che non possiamo parlare altro che di una sussidiarietà,

Se consideriamo l'etimologia della parola «sussidiarietà», vediamo che viene dal latino e significa «aiutare». Questa dimensione di aiuto, in un'accezione appunto di sussidiarietà circolare, non si trasforma nell'aspetto degenerativo dell'assistenzialismo, ma credo che invece acquisisca quel valore di grande eticità sociale che è il protagonismo sociale. Penso che questo debba essere il vero significato di un intervento che dia la possibilità di sostenere le persone che Grazie, non solo i termini «dignità» e «sussidiarietà» a fondamento del contrasto alla povertà, ma anche quelli, abbastanza significativi, di «fragilità» e «vulnerabilità»

e propositiva, come attori e non da comparse, alla stessa vita politica. Mi sembra allora che il contrasto alla povertà, oltre ad avere una valenza squisitamente di ordine socio‑economico, vada ad inerire anche tematiche di ordine politico e di assetto

metaforicamente inteso come il prodotto di una moltiplicazione i cui fattori rappresentano il bene delle singole persone o dei gruppi. È sufficiente modificare uno dei fattori e il bene comune non esiste più,

tali da incentivare anche il ruolo del terzo settore nella coprogettualità delle nuove iniziative locali contro la povertà, utilizzando la rete dell'associazionismo per avvicinare le persone emarginate che, altrimenti, continuerebbero a non essere raggiunte dalle misure economiche e di inserimento sociale, nonché al fine di poter offrire una maggior qualità e capillarità dei servizi. È opportuno incoraggiare sia i servizi istituzionali a livello territoriale che le organizzazioni *non profit*. Un altro aspetto che mi è caro sottolineare è che fino ad oggi la famiglia ha rappresentato il più importante ammortizzatore del disagio sociale, senza ricevere gli adeguati sostegni. Bisogna partire, quindi, dalla famiglia come soggetto di interventi, secondo quanto richiamato anche dalla Costituzione: la promozione la promozione di serie politiche familiari è lo strumento che meglio può accompagnare azioni mirate alla rimozione delle cause di povertà e di esclusione sociale in Italia. In parallelo, vi è la necessità di realizzare un sistema di *welfare* che assicuri livelli unitari di prestazioni in tutto il territorio nazionale, senza disparità, sperequazioni e differenze.

della prima, per un problema di natura squisitamente politica. Mi piace ribadire tale concetto. La vice ministro Guerra ha esordito sostenendo che nel primo punto

M5S)*. L'idea che si sia alle dipendenze del popolo italiano, che ci ha eletto per affrontare i problemi con cui quotidianamente operai, lavoratori, cittadini, agricoltori, commercianti, funzionari e *middle class*, forse non è fatta propria da chi ritiene

risulta capace di dividere? È una nozione su cui lo stesso Rodotà - un nome cui magari molti sono legati - ha impegnato tanti dei suoi ultimi studi. Rodotà ha presentato la sua riflessione sul diritto di esistenza come l'equivalente passato del diritto al reddito minimo garantito, del diritto di cittadinanza o comunque del diritto di dignità, che permetterebbe - come

partecipazione ad un contesto che insieme valorizza il sé sia a livello individuale sia soprattutto a livello sociale. Infatti, attraverso tale riconoscimento il gruppo si fa carico della singola individualità. La senatrice Bencini ha poc'anzi concluso il suo intervento riprendendo uno *slogan* che mi piace ripetere in quest'Aula: nessuno deve rimanere indietro. si possa permettere a tutti di non essere marginalizzati, di non essere isolati o dimenticati,

privilegi a cui non è disposta a derogare, giacché quando si ha un privilegio difficilmente lo si cede), oggi siamo chiamati ad operare quello sforzo di solidarietà per cui chi è rimasto indietro - e in Italia sono tanti possa capire che chi è avanti si sta fermando. Prima sono stati citati Stiglitz e Krugman, che in molti loro studi (non soltanto quelli più recenti) hanno evidenziato come in società patologicamente malate si registra un dato complessivo per cui il famoso PIL decrescerebbe e nel contempo le distanze sociali, economiche e culturali tra chi è sopra e chi è sotto si dilaterebbero. Noi abbiamo un'idea di comunità che è del tutto diversa e se questo ci porta alla divisione (vorrei che il Governo ne prendesse consapevolezza), divisione sarà, perché noi siamo per un'idea di comunità in cui tutti possano essere inclusi e non a parole, ma nei fatti. Proprio nei fatti chiediamo con insistenza che in queste Aule, che anche alla Camera stiamo lavorando in quel senso, si possa finalmente riconoscere l'eguale diritto di chi (e mi rivolgo alla senatrice della Lega che ha ricordato il suo passato di operaia), di operaia), pur non avendo un'estrazione sociale importante, possa sentirsi a tutto tondo, a pieno diritto,

dimostra che di ascolto forse non tutti sono capaci, perché non lo vogliono. Presidente, signora rappresentante del Governo, quando il Governo Berlusconi avviò la propria attività e avvertì l'approssimarsi di quella tempesta perfetta che avrebbe poi generato il lungo tempo di crisi in cui ancora siamo immersi, ritenne opportuna una riflessione ampiamente partecipata intorno al nostro modello sociale. I vincoli di finanza pubblica che dovevano necessariamente essere assunti avrebbero cioè potuto rappresentare una straordinaria opportunità per ripensare il nostro modello di protezione e di sicurezza sociale in funzione di una sua maggiore sostenibilità, non solo dal punto di vista finanziario, ma ancor più dal punto di vista della capacità effettiva di inclusione allora quella larga consultazione, con un metodo mutuato dall'Unione europea: prima un libro verde, infine la redazione di un libro bianco intitolato «La vita buona nella società attiva», frutto della collaborazione di circa 1.000 soggetti, tra di essi 100 rappresentativi di organizzazioni di vario genere, dalle associazioni etiche agli interessi organizzati. Credo si possa dire che quel libro bianco, come si registrò poi nel dibattito parlamentare che lo accompagnò, fu l'espressione non di una maggioranza parlamentare contingente, ma di convinzioni largamente condivise, perché la definizione del nostro modello sociale non può non collocarsi nella stessa Costituzione materiale che sostiene la stessa Costituzione formale. Quella larga condivisione riguardò soprattutto tre criteri, in base ai quali procedere ad un'intensa riorganizzazione delle sparse funzioni di protezione e di sicurezza sociale. I tre criteri individuati

non dell'individuo, perché nella nostra cultura, nella cultura della nostra tradizione, preferiamo parlare di persona, in quanto entità naturalmente vocata alla relazione con gli altri. La centralità della persona induce proprio a quei tre parametri e a rimuovere quei vizi di autoreferenzialità e di assistenzialismo insistito, che hanno caratterizzato frequentemente il nostro modello sociale. «Prevenzione» significa anche provvedere a che la persona, lungo tutto l'arco e in ogni fase della vita, possa essere messa nella condizione di provvedere alla propria autosufficienza, affinché non si determinino condizioni di bisogno o di dipendenza nella fase successiva. «Appropriatezza» significa integrare le funzioni:

arrivando ad immaginare un unico fondo nazionale, in cui far affluire anche risorse centrali, come quelle dedicate all'indennità di accompagnamento,

che il federalismo fiscale ha disegnato - i fabbisogni *standard* per le municipalità e i costi *standard* per i nostri servizi socio‑sanitari nei territori che consentano parità di opportunità per ciascuno dei tanti luoghi in cui si articolano le funzioni istituzionali e si organizzano le capacità sociali. Il caso della povertà e della povertà assoluta è straordinariamente emblematico a questo proposito. Della povertà assoluta abbiamo parlato: non confondiamola con la più ampia dimensione della povertà relativa, che è un utile indicatore per quanto riguarda la forbice che divide la nostra società e che serve ad effettuare politiche di riequilibrio da questo punto di vista. La povertà assoluta ci interessa perché rappresenta quell'area di bisogno estremo verso la quale dobbiamo concentrare le nostre energie, per prevenirla e per assorbirla quando si determina. La povertà assoluta non si identifica da Roma, attraverso una soglia di reddito, ma si identifica in prossimità, attraverso un complesso di indicatori soprattutto di carattere relazionale - infatti, spesso la solitudine è la vera e fondamentale fonte della povertà assoluta

quanto più possibile con altri enti locali, perché la microdimensione municipale evoca bisogni anche di integrazione e di razionalizzazione; ma soprattutto l'ente locale deve essere, a sua volta, scatenatore di vitalità sociale.

*social card*, di uno strumento che ha due caratteristiche: da un lato, quella di poter attrarre il dono, cioè di poter essere alimentata da quel dono che deve essere ricondotto dalla dimensione privata nella dimensione pubblica, perché il dono è già in sé strumento importante per realizzare capitale sociale, per costruire comunità, per assorbire i fenomeni di disagio sociale; dall'altra parte, la *social card* evoca strumenti di sostegno finanziario, ma anche di veicolazione di servizi, che devono essere devono essere a loro volta organizzati, gestiti, accompagnati al titolare del bisogno dalle nostre forme comunitarie. La *social card*, cioè, non è il modo di erogare freddamente un bene o un sostegno finanziario, ma è il modo con il quale le nostre organizzazioni sociali avvicinano la persona in condizioni di bisogno e la accompagnano ad una condizione di autosufficienza. È l'esperienza del banco alimentare, del banco farmaceutico; sono le infinite esperienze delle opere generose che hanno segnato questa Nazione ad indicarci la strada attraverso la quale isolare e assorbire le condizioni di bisogno. Per questa ragione, signor Presidente, signora rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, crediamo si debba procedere lungo quella strada, che si debba allargare l'esperienza, che soprattutto è stata ipotizzata per le città maggiori, nelle quali più si producono quei fenomeni di solitudine. In conclusione, voglio soltanto dire a coloro che ogni tanto parlano di modello nordico che quel modello è molto lontano dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura, perché è fatto di individui isolati che si confrontano direttamente con uno Stato anonimo, generoso anche nell'erogazione del sussidio, ma lontano e freddo, algido rispetto alla loro solitudine. *(Applausi del senatore* *Bitonci)*. Noi vogliamo restare ancorati alla nostra tradizione, alle nostre esperienze, a quelle esperienze delle opere generose che l'hanno costruita, che hanno fatto una Nazione prima ancora

vice ministro Guerra, colleghe senatrici e colleghi senatori, si è svolto questa mattina un dibattito a mio avviso importantissimo, importantissimo, che ha certamente significato la consapevolezza nostra, dei rappresentanti dei cittadini all'interno di questa istituzione,

È stato un dibattito ricco, con accenti e punti di vista diversi, ma fondamentale. Sappiamo che la pesante crisi economica nella quale ci troviamo, che ha visto precipitare in una condizione di povertà persone e famiglie, colpendo anche la classe media, rischia di aggravarsi producendo non solo un grande disagio materiale ma anche sfiducia e mancanza di speranza nel futuro. che questa sia una condizione oramai studiata e compresa, che ci obbliga da subito a trovare soluzioni concrete. firmatario il senatore Lepri, sono indicate le questioni di maggiore sofferenza ed anche le soluzioni. Noi apprezziamo le valutazioni e le considerazioni che il vice ministro Guerra ha indicato rispetto a questa mozione, ed è importante

accolgono, comprendono ed intervengono sui bisogni dei cittadini che versano in una condizione di povertà, che significa anche emarginazione e solitudine,

Permettetemi di fare una considerazione, che è stata fatta anche da molti colleghi e da molte colleghe: la condizione di povertà e di emarginazione, il rischio di povertà materiale in cui si trovano tante persone singole e tante famiglie, comportano altresì, come dicevo prima, un senso di sfiducia verso il futuro. La condizione

verso il futuro, che significa anche un'ulteriore e progressiva diminuzione dei consumi. Pensiamo

la frequentazione delle mense sociali veda sempre più numerosa la presenza di cittadini e cittadine fino a poco tempo fa, potevamo considerare appartenenti alla classe cosiddetta media, in una condizione cosiddetta normale. La povertà è una condizione che, nel nostro Paese, tocca fasce di popolazione che sino a qualche anno fa vivevano in una situazione di cosiddetta normalità. Ma la perdita del posto di lavoro, una malattia invalidante che colpisce un membro della famiglia,

nelle cronache quotidiane del nostro Paese situazioni di grande drammaticità. Tutto ciò non ha trovato in questi ultimi anni una risposta concreta ed incisiva, con l'attivazione di servizi che potessero essere almeno un sollievo per i disagi delle famiglie da parte degli enti locali, gravati, come sappiamo, da tagli drammatici sul Fondo delle politiche sociali, dai famosi tagli lineari, da tante questioni che hanno progressivamente costretto le amministrazioni a tagliare servizi essenziali di sostegno e di accompagnamento

aiuteremo i cittadini che oggi versano in uno stato di grande povertà, ma addirittura aggraveremo questa situazione. è stato ripetuto da molti - che non è soltanto una questione economica, ma in questo momento la questione economica appare essenziale. È evidente che, in un momento storico in cui le risorse diminuiscono, è necessario riprogettare in maniera diversa alcune tipologie di intervento. In questo momento nel nostro Paese sono presenti soggetti che tradizionalmente hanno contribuito negli anni a

vero, approfondito, puntuale con il mondo della cooperazione sociale, dell'associazionismo, del volontariato, i quali sono assolutamente consapevoli della drammatica condizione economica che vive il nostro Paese. Sono quelli i soggetti che hanno collaborato con i servizi pubblici e con gli enti locali, che negli anni Ottanta hanno progettato con il pubblico la qualità e l'innovazione delle politiche sociali nel nostro Paese. Credo che dobbiamo ridare dignità a questo rapporto, valorizzare e richiamare a protagonisti della progettazione gli operatori pubblici che lavorano nei settori dei servizi socio‑sanitari, perché essi sono la ricchezza, sono le gambe che fanno camminare ciò che nelle istituzioni

di un impegno vero e concreto delle istituzioni, ma dà il senso del pensiero che voglio rappresentare. È una frase di don Milani, il quale che fare parti uguali tra uguali è giustizia, fare parti uguali tra disuguali è somma ingiustizia.

Presidente, noi siamo contrari alla votazione per parti separate. Riteniamo che la mozione debba essere votata nella sua interezza.

più che il mantenimento del punto 1) in sé è proprio la motivazione con cui questo mantenimento è stato presentato, che ha voluto sottolineare una divisione di vedute, che non mi permette di accogliere la richiesta. Quindi confermo il parere contrario.

Tale votazione avverrà, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, a scrutinio segreto sulle seguenti liste di candidati formate su designazione dei Gruppi parlamentari.

Membri supplenti, senatori: Puppato, Lucherini, Verducci, De Pietro, Orellana, Amoruso, Fazzone, Munerato e Cervellini. I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Presidente. Se io questo caffè da cittadino abruzzese volessi pagarlo con le *royalty* che prendiamo, derivanti dal pessimo petrolio che abbiamo nei fondali marini dell'Adriatico,

C'è un pericolo di inquinamento nel Mediterraneo, derivante dalle attività connesse di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il rischio che tali attività comportano non è trascurabile e non può essere più sottovalutato e rinviabile, in quanto reca con sé l'enorme minaccia al patrimonio composto da riserve marine, coste pregiate ad alta vocazione turistica, pesca e cultura dell'ambiente. A poco più di due mesi dalla manifestazione di Pescara, in cui 40.000 persone sfilarono per dire no a "Ombrina" e no alla trasformazione dell'Abruzzo... *(Brusìo)*.

Mi permetto di tornare un po' indietro, perché è importante. Sono passati poco più di due mesi da una manifestazione in Pescara in cui 40.000 persone hanno sfilato per dire no al progetto "Ombrina Mare" e no alla trasformazione dell'Abruzzo, nota a tutti come Regione verde, in distretto minerario. Sia le associazioni che i comitati *green* che i cittadini sono più che mai uniti per ribadire le ragioni del loro no fermo e convinto alle trivellazioni, mentre dicono si a scelte ed alternative più ragionevoli. Ritengo che oggi il Senato, venendo finalmente incontro alle richieste provenienti dal territorio, dai cittadini e dalle associazioni, ma anche venendo incontro alle richieste degli onorevoli senatori del PdL (Dalì e altri, Marinello e altri), nonché degli onorevoli senatori del «PD meno elle» (Pezzopane e altri, Tomaselli e altri), che rispettivamente hanno presentato i disegni di legge nn. 222 e 460, possa facilitare, con un voto favorevole a questa mozione, il primo passo verso il riavvicinamento tra istituzioni e bisogni reali dei cittadini.

l'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare; restituiscono l'efficacia ai titoli abilitativi rilasciati prima dell'agosto 2010; salvano in modo retroattivo i procedimenti antecedenti all'agosto 2010, tra i quali il progetto di coltivazione del giacimento "Ombrina Mare". Ripeto: lo salvano. Tutte queste modifiche al codice dell'ambiente non sono mai state discusse dal Parlamento, ma sono il risultato della questione di fiducia posta dal precedente Governo all'interno del decreto-legge n. 83 del 2012, che è stato così approvato, estromettendo, come sempre, il Parlamento dalla possibilità di emendarlo. Non è neanche il caso di ricordare l'imbarazzante lettera di ringraziamento inviata dalla Medoilgas Italia SpA al ministro Clini. È invece opportuno oggi sottolineare che l'area marina in cui si sviluppa il progetto "Ombrina Mare" dista solo 6 chilometri (non miglia, ma chilometri) dal Parco nazionale della Costa teatina, così come disposto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione Abruzzo interessata. Deve sottolinearsi che il territorio della costa teatina e, in generale, quello dell'intero Abruzzo sono caratterizzati dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva ed apprezzata. Tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse. Lo sviluppo del progetto "Ombrina Mare 2" certamente comprometterebbe la realizzazione di un sistema regionale integrato "mare-montagna", di sviluppo economico e sociale sostenibile, su cui la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive, le associazioni dei cittadini sono fortemente orientati, motivo per cui, in sede di valutazione di impatto ambientale sono state presentate numerosissime osservazioni e obiezioni anche da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dalle realtà territoriali portatrici di interessi. Non può tacersi che, in base alla normativa vigente, la commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale aveva espresso sul progetto in questione parere negativo e che, dalla data di preavviso di rigetto della VIA, comunicata alla Medoilgas Italia SpA sul progetto "Ombrina Mare 2", il Ministero non ha mai adottato - ripeto mai - il provvedimento di diniego, nonostante non sussistesse alcun impedimento formale. L'ingiustificata mancata adozione definitiva del provvedimento di reiezione della VIA ha permesso il riavvio dello stesso procedimento di VIA e, in applicazione della nuova disciplina, la commissione tecnica di verifica ha magicamente espresso parere positivo al progetto. Si continua comunque erroneamente a ritenere che si possano risolvere le questioni abbreviandone i tempi e l'*iter* o convincendo le popolazioni ad abbandonare le opposizioni locali, nate da semplici ma giustificate paure, o anche dalla mancanza di dialogo con le amministrazioni. Probabilmente, l'accesso alle informazioni in materia di energia e ambiente è proprio il punto sul quale l'Italia da sempre manca di strategia e di visione. Siamo il Paese dove si trivella con il *fracking* da decenni e nessuno lo sa; dove si muore di inquinamento a Taranto ma si ritarda la pubblicazione dei dati scientifici che lo dimostrano. Siamo il Paese dove, per sapere chi sono i personaggi politici favorevoli a petrolio o carbone occorre una campagna di Greenpeace. Perseveriamo nell'errore senza renderci conto del potenziale espresso dal nostro Paese in tema di sviluppo della *green and white economy*, che attraversano e innovano anche i settori più maturi della nostra economia. Troppo spesso ci si dimentica di alcuni strumenti che potrebbero realmente cambiare il sistema energetico nazionale, creando tra l'altro ricchezza e occupazione per le piccole e medie imprese e per le famiglie senza privilegiare gli interessi di pochissimi a scapito di tutti gli altri. Con questi presupposti programmare il futuro è impossibile. L'Italia, praticamente, rinuncia a farlo. Ebbene, ad oggi, i parlamentari di ogni schieramento, compresi alcuni attuali componenti del Governo, quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Giovanni Legnini, firmatario assieme ad altri di una proposta di legge in merito, hanno dato vita a numerose iniziative legislative riguardo alle modifiche da apportare all'articolo 35 del decreto n. 83 del giugno 2012, iniziative iniziative tutte volte ad annullarne, limitarne o, quantomeno, modificarne gli effetti. Per tutti questi motivi, noi oggi chiediamo un voto positivo sulla mozione n. 39, il cui assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare il benedetto articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ripristinare il divieto di attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia, anche per i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Il secondo punto chiede di sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già depositati presso i due rami del Parlamento. Il terzo punto chiede la revoca del provvedimento di accoglimento della VIA contenuto nel parere n. 1192 del 3 aprile 2013. chiede la revoca dei titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 128 del 2010, e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia di tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi. Il quinto punto sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo, n. 152 del 2006, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

Ciò che sta avvenendo nell'alto Adriatico indubbiamente preoccupa le popolazioni e i territori. La regolamentazione si è succeduta nel tempo, ma noi vorremmo mantenere molto rigida la tutela dell'alto Adriatico. Il Mediterraneo, lo sappiamo, è di per sé un mare chiuso,

alcunché, se non da parte dei fotografi autorizzati nelle loro apposite tribune.